Sbarbati, che chiede notizie in merito alla chiusura dei corsi di laurea in Lingue e comunicazione e operatore culturale per il turismo dell'Università degli studi di Cagliari, il rettore, premettendo che non è stata data alcuna comunicazione del tenore riportato nell'interrogazione, come pure non è pervenuta agli uffici amministrativi o agli organi accademici dell'ateneo alcuna segnalazione in merito ad irregolarità dell'attività didattica o delle procedure di immatricolazione per i menzionati corsi, riferisce quanto segue. Per il prossimo anno accademico 2009-2010, allo stato, non si è deliberato in merito alla trasformazione o modifica dei suddetti corsi. In ogni caso le decisioni che l'ateneo assumerà saranno conformi alle norme che disciplinano la materia e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del decreto nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, che l'Università garantisca agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. Nel corrente anno accademico, il corso di laurea in lingue e comunicazione, classe 14, della facoltà di lingue e letterature straniere, istituito ai sensi del decreto (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), nell'anno accademico 2005-2006 è stato regolarmente attivato nel rispetto delle disposizioni ministeriali e successivamente inserito nel Manifesto generale degli studi pubblicato il 1° luglio 2008. Le immatricolazioni al primo anno e le iscrizioni agli anni successivi sono avvenute regolarmente secondo quanto disposto nel regolamento didattico di ateneo e nel Manifesto generale degli studi del corrente anno accademico: risultano iscritti al primo anno di corso 191 studenti, non vi è stata alcuna sospensione delle lezioni e gli esami, distinti in due semestralità, si svolgono regolarmente. Si precisa, inoltre, che il corso di laurea in operatore culturale per il turismo, classe 39, istituito nell'anno accademico 2004-2005 ai sensi del citato decreto a seguito dell'applicazione del decreto ministeriale n. 270 del 2004, è stato trasformato nel corso di laurea in scienze del turismo, classe L-15, interfacoltà, tra economia, giurisprudenza e lettere e filosofia. La suddetta trasformazione ha comportato per il 2008-2009 l'attivazione del solo primo anno del citato corso in scienze del turismo, al quale risultano iscritti 90 studenti, contestualmente alla disattivazione del primo anno di quello in operatore culturale per il turismo e l'attivazione soltanto del secondo e terzo anno di quest'ultimo, ormai ad esaurimento, per 468 studenti. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dalle suddette disposizioni, è stata garantita agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, consentendo ai medesimi di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. Per quanto riguarda l'offerta didattica del corso di laurea in operatore culturale, si fa presente che vengono garantiti gli insegnamenti relativi al secondo e al terzo anno, mediante l'attivazione di insegnamenti specifici, oppure attraverso insegnamenti relativi ai corsi attivati decreto ministeriale n 270 del 2004, nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia che, formalmente o sostanzialmente, coincidono con gli insegnamenti del suddetto corso di operatore culturale per il turismo.

Se risponde al vero quanto lei ha oggi riportato in quest'Aula, come frutto di informazione da parte dell'ufficio del Ministero - terminale dell'informazione il rettore della stessa università - credo bisognerà fare un'indagine precisa - e per quanto mi riguarda la farò sicuramente - per verificare se quanto egli ha fornito a

Credo sia un atto dovuto, anche perché le segnalazioni sono plurali e credo che il dover garantire a studenti che hanno contratto con l'università un patto patto specifico di impegno - altrettanto specifico e reciproco - rispetto ad un percorso di studi che inizia e deve avere una fine e delle garanzie (ed anche dei supporti didattici specifici e delle attrezzature altrettanto specifiche),

secondo volontà o decisioni che non hanno né capo né coda e quantomeno non sono supportate né suffragate da un contatto con il mondo studentesco, il mondo accademico e la realtà sociale in cui l'università comunque è inserita. Se parliamo di università, ogni università ha un suo retroterra, un suo retroterra, che è fatto di cultura antropologica, sociale, storica ed anche economica ed a questo contesto ci si deve riferire nel momento in cui si istituisce o si abolisce un corso di laurea.

e non certo lo spirito culturale che dovrebbe animare un Ministero che guarda all'università come il fulcro ed il motore di una sapienza *in fieri*, che il nostro Paese deve conquistare giorno per giorno per essere capace di competere a livello internazionale. La nostra capacità di competizione richiama semplicemente ed esclusivamente ad una competenza, ad una specificità e ad una capacità culturale e creativa che soltanto università libere ed aperte,

a percorsi che devono essere possibili per tutti, perché pari opportunità per i capaci e meritevoli e anche solidarietà il nostro Stato li garantisce attraverso la Costituzione repubblicana.

occorre premettere che la legge n. 410 del 2001, che ha dato avvio al processo dì dismissione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso lo strumento della cartolarizzazione, all'articolo 2, comma 2, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca semestralmente al Parlamento in merito ai risultati economico-finanziari conseguiti. In linea con tali disposizioni, l'amministrazione ha avviato un processo di monitoraggio dedicato alle dismissioni e ai proventi derivanti dalle operazioni in questione, anche a tutela dei portatori dei titoli, come previsto dall'articolo 7 dei decreti 18 dicembre 2001 e 21 novembre 2002, relativi rispettivamente alla prima e alla seconda operazione di cartolarizzazione. Sulla base di un *business plan* economico, i proventi derivanti dalle vendite hanno consentito alla SCIP il rimborso del debito contratto sui mercati con l'emissione dei titoli. Per quanto riguarda le operazioni effettuate dal Governo nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e controllo sull'ente gestore, si precisa che il controllo esercitato ha la finalità di verificare che gli impegni assunti dall'ente gestore nell'ambito dell'apposito contratto siano adempiuti secondo i criteri stabiliti. In proposito, si richiama l'allegato 4 ai decreti 30 novembre 2001 e 21 novembre 2002, relativamente alla prima e seconda operazione di cartolarizzazione, che sinteticamente riepiloga gli impegni e le obbligazioni a carico dei gestori. Inoltre, l'articolo 10 del citato contratto consente all'ente di delegare una parte delle attività di natura squisitamente gestoria ad apposite società, esclusa la rappresentanza nell'atto di compravendita, che l'ente stipulava in nome e per conto della SCIP. Tale previsione contrattuale ha consentito la prosecuzione dei contratti di gestione in essere, stipulati tra taluni enti e le società di gestione prima dell'avvio delle operazioni di cartolarizzazione, riguardando attività quali la manutenzione, la riscossione dei canoni, la regolarizzazione catastale e così via, il cui contenuto non strategico, ma squisitamente operativo, non poteva essere svolto direttamente dall'ente, data la natura istituzionale del medesimo, nonché la non specifica professionalità in materia immobiliare. Prima della procedura di liquidazione, la SCIP ha effettuato una puntuale *due diligence* sul portafoglio residuo, tesa a conoscere in modo capillare le situazioni di incaglio che hanno generato il contenzioso, soprattutto con riguardo alle posizioni debitorie da parte degli inquilini titolari di regolare contratto di locazione, ma non in regola con i pagamenti, o con contratti scaduti. Si precisa, inoltre, che il trasferimento dei beni dagli enti alla SCIP ha congelato lo *status* giuridico-fattuale del patrimonio e, pertanto, come rilevabile dai decreti e dai contratti di gestione stipulati, agli enti non era consentito provvedere al rinnovo dei contratti scaduti, ad eccezione del portafoglio commerciale, nei modi e nelle circostanze previste dal decreto di trasferimento. In forza di quanto previsto dai contratti di gestione, con particolare riguardo all'impegno sottoscritto dagli enti di provvedere, ai sensi delle disposizioni vigenti, ma con la cura e l'attenzione del buon del buon *pater familias*, sono state poste in essere tutte le procedure di conciliazione con gli inquilini o con le loro rappresentanze, tese a risolvere quelle situazioni legittimamente sanabili, al fine di consentire ai medesimi l'esercizio dell'opzione d'acquisto, secondo quanto prescritto dall'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 410 del 2001. Tale procedura ha consentito, nella maggior parte dei casi, di procedere alla vendita dei beni ai conduttori medesimi, tranne in limitate situazioni, che non sono state risolte a causa di problematiche attinenti l'effettiva titolarità del diritto all'acquisto. Con riferimento ai diritti spettanti agli aventi diritto, l'articolo 43-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, dispone che gli stessi sono fatti salvi. Tale principio di salvaguardia era previsto anche nella legge n. 410 del 2001. Pertanto, il diritto all'acquisto del bene, sia in forma individuale che in forma collettiva, ove ricorrano i requisiti previsti dal menzionato comma 6, è inviolato e l'ente proprietario provvederà secondo la propria programmazione di vendita ad alienare alle medesime condizioni economiche richiamate dalla legge n. 410 del 2001, ivi compresa l'applicazione degli sconti *ex lege* e del riconoscimento dell'eventuale ulteriore coefficiente di abbattimento previsto dalla legge n. 104 del 2004, riconosciuti a quanti avessero manifestato la volontà d'acquisto del bene entro l'ottobre 2001, mediante l'invio di apposita raccomandata. Per quanto riguarda, infine, la regolarizzazione contrattuale delle posizioni ancora non risolte, è indubbio che, stante l'esercizio da parte dell'ente della piena titolarità del bene, tale processo sarà agevolato ove ricorrano le circostanze che la disciplina generale in materia di locazione prevede che si concilino con il riconoscimento del diritto d'opzione contemplato dall'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 410. Pertanto, conclusivamente si può affermare che l'intendimento del legislatore è quello di dare continuità al processo di alienazione del patrimonio degli enti, avviato ancor prima delle operazioni di cartolarizzazione, assecondando le aspettative di coloro che legittimamente vantano il diritto d'acquisto degli immobili ad essi locati.

*(PdL)*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Pizza per la risposta articolata e precisa che segnala una seria attenzione ai quesiti che ho posto alla pubblica amministrazione.

che riguarda sostanzialmente la cessione di beni o di strutture dello Stato (in particolare appartamenti) a coloro che regolarmente vi abitavano o vi abitano,

disciplinato un argomento già preso in considerazione dall'INPS e dagli altri organi di previdenza, oggi, nel 2009, veda ancora delle pratiche non risolte.

Come è possibile che nel 2008 il Governo sia costretto, con il citato articolo 43*-bis*, a sollecitare questi organi a provvedere perché in breve si realizzino

il quale è anche sotto inchiesta. Ringrazio quindi il Governo per la serietà con la quale è venuto a riferire

Governo ha citato e scritto «intenda assumere al fine di: a) definire il contenzioso immobiliare in atto, attraverso la proposizione di specifiche soluzioni transattive», come recita lo stesso articolo, raggiungere il bonario componimento con gli ex inquilini e inquilini ormai prossimi a intraprendere azioni giudiziarie». Infatti, se gli inquilini hanno intenzione di intraprendere azioni giudiziarie evidentemente ve ne sono le motivazioni; altrimenti nessun inquilino a cui la legge attribuisce la facoltà di ricevere in cessione l'appartamento che abita si sogna di innescare un procedimento giudiziario. Ed infine: «se e quali misure il Governo adotterà per tutelare e salvaguardare i diritti di tutti i conduttori, sia di quelli che hanno esercitato la prelazione nell'esito positivo della vendita, sia di quelli che sono stati impossibilitati all'esercizio del diritto di opzione e hanno diritto al rinnovo del contratto». La speranza è che questo Governo,

prevedeva che, in attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi, il mandato quadriennale del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dell'INAlL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA venisse prorogato fino al 28 luglio 2008, termine di scadenza dei consigli di amministrazione degli istituti medesimi. Successivamente è stato disposto, con decreti interministeriali in data 11 settembre 2008, il commissariamento dei predetti enti, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere da *a)* a *c)* della legge n. 133 del 2008, che prevede l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusi gli enti pubblici non economici, secondo princìpi di efficienza, razionalità ed economicità, in modo da assicurare la complessiva riduzione delle relative spese di funzionamento. La necessità di procedere ad un'istruttoria supplementare, ai fini della corretta ponderazione dei parametri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la ricostituzione dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli istituti citati, ha determinato il conferimento ai commissari straordinari delle competenze spettanti ai suddetti organismi. Al riguardo, si rappresenta che con decreti adottati in data 2 gennaio 2009 sono stati ricostituiti i predetti Consigli di indirizzo e vigilanza. Inoltre, con decreti interministeriali, in data 27 marzo 2009, i commissari straordinari degli enti previdenziali pubblici sono stati confermati nell'incarico fino al completamento del processo di riorganizzazione previsto dal citato decreto legge n. Per quanto concerne i rilievi di cui all'atto parlamentare, inerenti il bilancio dell'INPS, sono in grado di informare che il bilancio consuntivo dell'istituto relativo all'anno 2007, predisposto dal consiglio di amministrazione

L'assestamento al bilancio preventivo 2008, approvato dal commissario straordinario con determinazione n. 85 del 20 novembre 2008, è stato approvato in via definitiva dal commissario straordinario del Consiglio di indirizzo Il bilancio preventivo per l'anno 2009, predisposto dal commissario straordinario con determinazione n. 87 del 24 novembre 2008, è stato approvato in via definitiva dal commissario straordinario del Consiglio di indirizzo

conseguenti alle disposizioni di cui alla legge finanziaria per il 2009, ed in particolare alle previste riduzioni dei trasferimenti statali all'INPS (articolo 2, comma 26), ai fini di poter procedere ad eventuali correttivi, occorrerà preventivamente valutare, nel concreto, gli effetti di tali disposizioni con riferimento all'andamento, nell'anno, delle relative gestioni.

vi sono tre questioni che rimangono del tutto insolute. La prima riguarda la nomina dei consigli di amministrazione: di un *vulnus* poco rilevante rispetto al buon funzionamento e all'assetto degli organi degli enti previdenziali. Il fatto, tra l'altro, che nel frattempo si sia proceduto all'approvazione della nota di variazione del bilancio, poi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, ha fatto sì che la figura del controllore coincidesse con quella del controllato. Credo che questo metterà a rischio il giudizio che la Commissione di vigilanza degli enti previdenziali dovrà dare sulla correttezza degli atti amministrativi che si sono svolti in questo periodo. Credo poi sia abbastanza singolare che si sia motivata la mancata nomina dei Consigli di amministrazione con una generica impossibilità invocata dal Governo: sarebbe utile sapere qual è l'impossibilità che il Governo invoca per prorogare per ben un anno e mezzo e per commissariare per ben un anno e mezzo dalla loro naturale scadenza i Consigli di amministrazione.

in ordine ai conti pubblici, di risparmi attesi dal bilancio dello Stato. Con tre miliardi e mezzo, in questi tempi in cui discutiamo se 200 milioni siano la cifra giusta per la ricostruzione faraonica dell'Abruzzo, ne potremmo ricostruire diverse di città come L'Aquila. Eppure, questo percorso non lo si fa e nemmeno si mettono all'ordine del giorno i provvedimenti che ne erano propedeutici, ad esempio la presentazione del piano industriale previsto dalla legge del 2007 lasciata dal Governo Prodi, che doveva individuare le modalità in cui questa riorganizzazione sarebbe stata realizzata. Credo che questo modo di procedere non sia accettabile dal punto di vista della correttezza della gestione della cosa pubblica e dei grandi enti previdenziali, che - ricordo - garantiscono la previdenza per la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti del nostro Paese. Ricordo, inoltre,

credo sia convenuto e riconosciuto da tutti che la questione della sicurezza sul lavoro è una delle priorità nel nostro Paese.

si allentino l'interesse e l'attenzione sulle questioni della sicurezza sul lavoro. C'è poi un altro aspetto che speravo di trovare nella risposta del Governo e che non ho trovato. Il Governo trasferisce

del fondo lavoratori dipendenti, che andrà in rosso, e quindi l'attivo si azzererà. Il passivo sarà ripianato con il fondo lavoratori parasubordinati, cioè quello per i giovani è inaccettabile che queste platee di assicurati, per i quali non si prevede nel tempo un futuro assicurativo degno di questo nome (tutti ci stiamo esercitando per vedere come far recuperare questa parte di svantaggio che i giovani accumulano per effetto dei cosiddetti rapporti di lavoro flessibili nella prima parte della vita lavorativa), vengano ulteriormente penalizzate dalle manovre di bilancio che si fanno nell'INPS trasferendo a loro carico l'azzeramento dell'attivo del fondo lavoratori dipendenti.

una preoccupazione: non è un caso che non si sia proceduto al rinnovo dei consigli d'amministrazione, prorogati ulteriormente fino a luglio, e che la risposta che il Ministro ha dato qualche giorno fa in Commissione di vigilanza sugli enti previdenziali faccia prefigurare che addirittura quella proroga è già adesso, nei fatti, un'altra proroga. Si vuole azzerare il sistema di *governance* in termini di autonomia degli enti,

quanto previsto anche dallo Statuto dei diritti dei lavoratori, che prevede che siano le parti sociali ad amministrare i contributi che provengono dalla devoluzione delle partecipazioni partecipazioni delle imprese e dei lavoratori alla costruzione della loro spesa e dei loro benefici previdenziali. Se si altera questo meccanismo

La senatrice Mongiello solleva l'attenzione sulla situazione occupazionale di una società, la Servizi Informatici srl, con sede a San Severo di Foggia, che svolge attività di acquisizione documenti, gestione *call-center* e centralino, gestione protocollo e spedizioni per conto della Banca Apuleia SpA, con una consistenza organica, al gennaio del corrente anno, pari a 18 unità lavorative. Fino al mese di dicembre 2008 la società in argomento ha operato anche per conto della Banca popolare di Bari, istituto che, insieme alla Banca Apuleia su citata, figura tra i proprietari della società medesima, con quote pari al 20 per cento Le vicende evidenziate nell'atto parlamentare inerenti l'avvenuto licenziamento di alcune lavoratrici, secondo le informazioni fornite dalla competente direzione provinciale del lavoro, sarebbero da ricondurre al mancato rinnovo del contratto di fornitura servizi da parte della Banca popolare di Bari, con conseguente esubero delle lavoratrici addette proprio ai servizi forniti al citato istituto bancario. In via generale, vorrei ricordare, con riferimento a presunti comportamenti antisindacali da parte del datore di lavoro, adombrati nell'atto ispettivo, che, come è noto, l'ordinamento qualifica come nulli tutti i patti e gli atti, tra cui i licenziamenti, connaturati da finalità discriminatoria ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 300 del 1970, determinata dalla affiliazione sindacale del lavoratore, dalla sua partecipazione ad attività sindacale o ad uno sciopero, o basati sulla discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso. Avverso gli stessi il lavoratore può agire in giudizio individualmente. Con riferimento, inoltre, agli atti volti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale è previsto lo speciale strumento di tutela di cui all'articolo 28 della medesima legge. In particolare, la predetta norma stabilisce che la mancata ottemperanza, da parte del datore, al decreto del giudice che ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti conseguenti è perseguita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Per quanto concerne il profilo relativo alla generale situazione occupazionale della provincia di Foggia,

consegnerò alla senatrice stessa le tabelle fornite dalla Regione Puglia che evidenziano, particolarmente, i dati inerenti l'occupazione femminile. In conclusione, vorrei rassicurare la senatrice in ordine all'attenzione prestata dall'amministrazione che rappresento verso le vicende quali quella all'attenzione, nelle quali potrebbe configurarsi la violazione dei diritti di libertà e di espressione sanciti a livello costituzionale, impegnandomi, nel contempo, a fornire direttamente alla senatrice le eventuali ulteriori notizie sulla vicenda in parola.

nel mancato rinnovo, incappano nella norma del licenziamento. È ovvio che tutte le lavoratrici potranno poi avvalersi degli strumenti legislativi - di questo ne siamo consapevoli

tutela dello stesso *parterre* di lavoratrici, che ancora una volta vengono penalizzate. Se a questo uniamo il fatto che in una particolare provincia e in un particolare momento come quello attuale si verificano tutta una serie di episodi, allora comprendiamo come sia difficile per queste donne

nel settore degli elettrodomestici bianchi con stabilimenti ubicati sul territorio nazionale (Marche, Umbria e Emilia-Romagna) e all'estero (Ucraina, Finlandia e Svezia). Da qualche anno, a causa della complessità del mercato degli elettrodomestici, l'azienda ha registrato un calo netto delle vendite. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 ottobre 2008, la società Antonio Merloni è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta legge Marzano). Nell'ambito di tale procedura è stata prevista, per un numero complessivo di 3.105 lavoratori,

La procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alle società controllate dal gruppo: Antonio Merloni Cylinder & Tanks Srl, Tecnogas SpA ed Elmarc SpA, rispettivamente in data 22 ottobre 2008, 7 novembre 2008 e 25 novembre 2008. I commissari preposti, avendo rilevato la necessità di nuovi finanziamenti per proseguire la produzione, hanno intrapreso l'*iter* per ottenere la garanzia dello Stato sul finanziamento bancario. A seguito della decisione favorevole della Commissione europea del 28 gennaio 2009, i commissari hanno proceduto, previa verifica e trattativa con le banche, ad individuare gli istituti di credito, interessati a concedere il finanziamento. Si evidenzia, inoltre, che con provvedimenti, emanati dalla competente Direzione generale del Ministero, del 25 marzo 2009 e del 15 aprile 2009, i commissari sono stati autorizzati alla definizione del contratto di finanziamento, per il quale è stata ravvisata la necessità della garanzia dello Stato, con Banca Marche SpA, per un importo complessivo sino a 30 milioni di euro. Al riguardo, si precisa che presso il Ministero dell'economia è in corso l'*iter* istruttorio per la concessione della prevista garanzia da parte dello Stato. Si segnala, inoltre, che in data 6 aprile 2009, a seguito di un sondaggio del mercato, effettuato attraverso la raccolta delle manifestazioni di interesse, è stato depositato il programma di cessione delle società in amministrazione straordinaria: Antonio Merloni SpA, Antonio Merloni Cylinder & Tanks Srl, Tecnogas SpA ed Elmarc SpA, attualmente in fase istruttoria. Si fa, altresì, presente che il Ministero dello sviluppo economico ha costituito un gruppo di lavoro tecnico finalizzato all'individuazione di programmi di riqualificazione e reindustrializzazione dei territori interessati dalle attività del gruppo Antonio Il 17 aprile scorso ad Ancona si è svolto un incontro, al quale hanno partecipato i rappresentati del Ministero e i rappresentanti della Regione Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, per verificare gli sviluppi della situazione del gruppo. Nel corso di tale incontro, è stato manifestato l'impegno a sostenere l'accordo di programma presentato dalle Regioni e a consolidare gli effetti produttivi ed occupazionali in esso contenuti. Al riguardo, si precisa che in relazione all'accordo di programma, verrà stipulato un preliminare protocollo di intesa, finalizzato a raccogliere un più ampio consenso di tutti soggetti interessati al rilancio dell'area coinvolta dalla crisi industriale della società. Il Ministero dello sviluppo economico, anche in questa occasione, ha confermato l'impegno a seguire con la massima attenzione le prospettive di rilancio del gruppo.

*(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il Governo, oggi rappresentato dal sottosegretario Romani, per aver risposto alla mia interpellanza, anche se vorrei sottolineare che sono passati ben sette mesi dalla data in cui è stata presentata, pur trattandosi di un atto con procedura abbreviata e, in particolare, di un'interpellanza con con procedura d'urgenza. All'epoca non si aveva ancora notizia ufficiale della proclamazione dello stato di crisi della Antonio Merloni SpA ai sensi della legge Marzano. Quindi, il Sottosegretario ha chiaramente evidenziato ed esposto il percorso intrapreso dal Governo in questi mesi per addivenire alla risoluzione della crisi aziendale. Tale percorso è stato composto da atti e provvedimenti di cui ero per la gran parte a conoscenza. Vorrei però ribadire la forte preoccupazione che la popolazione e le istituzioni dell'Umbria e delle Marche nutrono in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali e in merito al rilancio dell'attività economica nelle zone in cui sono ubicati i siti produttivi dell'azienda Antonio Merloni SpA, che potrebbero comunque subire conseguenze legate all'attuale crisi che ancora non è risolta, tenendo conto del fatto che essa si inserisce all'interno di una recessione globale che ha effetti anche sull'economia nazionale. Ricordo che l'azienda occupa circa 7.700 lavoratori (compreso l'indotto) nelle province di Ancona, Perugia e Reggio Emilia e che da ottobre a gennaio sono stati coinvolti nella cassa integrazione circa 960 operai nel solo stabilimento di Nocera Umbra, che fa parte della Regione che io rappresento. come ci ha riferito il Sottosegretario, il Governo ha concesso la garanzia dello Stato in relazione proprio all'amministrazione straordinaria dell'azienda, ora importante che nel più breve tempo possibile siano messe in atto tutte le misure idonee a sostenere i livelli occupazionali (quindi il reddito dei lavoratori)

alla configurazione geografica dei territori della zona appenninica, dove altre attività economiche non hanno un'importanza e una rilevanza pari a quelle dell'azienda Antonio Merloni. ragione, ritengo che in questa sede sia opportuno sollecitare la sottoscrizione da parte del Governo dell'accordo di programma già all'esame del Ministero (come è stato riferito), che contiene la previsione di impegni da parte del Governo e delle Regioni

per dare certezza a tutte le situazioni sospese, sia occupazionali che produttive. Teniamo conto del fatto che in questo momento i lavoratori stanno andando a lavorare in un'azienda che, soprattutto nel territorio umbro e marchigiano, chiude e apre a singhiozzo. e apre a singhiozzo. Infine, in considerazione del fatto che l'attuale crisi sta gravando pesantemente su famiglie e imprese che sono residenti in territori che sono

Il giudizio positivo sull'attività e sul ruolo della Fondazione Bordoni nel biennio 2007-2008 è condivisibile e condiviso, così come l'apprezzamento per l'azione svolta dal presidente, professor Decina, e dal direttore generale, professor Sassano, che ne hanno assicurato la guida. Ciò premesso, si ricorda che proprio su iniziativa del presidente Decina e su impulso del Ministro delle comunicazioni del precedente Governo si è proceduto a un significativo mutamento dello Statuto della fondazione stessa. Sulla base del precedente Statuto, la *governance* della Fondazione era largamente espressa dagli operatori privati e dalle società manifatturiere che, oltre a detenere una larga maggioranza nel consiglio di amministrazione, ne erano anche i finanziatori. Tale situazione, in considerazione del ruolo terzo che deve essere assicurato dalla Fondazione come istituzione di alta cultura riconosciuta dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, avente lo scopo di effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici ed applicativi nelle materie delle telecomunicazioni, dell'informatica, dell'elettronica e dei servizi multimediali in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica, avrebbe potuto determinare una sovrapposizione di interessi. Si è quindi proceduto a un mutamento dello Statuto che vede un consiglio di amministrazione di nomina pubblica, composto da sette componenti: uno indicato dal Presidente del Consiglio, due su cui deve convergere il parere del Presidente dell'AGCOM, e gli altri quattro designati dal Ministro dello sviluppo economico. I componenti sono tutti nominati dallo stesso Ministro e sono stati individuati in base alla loro indiscussa competenza tecnica e/o giuridica. Secondo il nuovo Statuto i rappresentanti dei soci privati, operatori di TLC e società manifatturiere, danno vita al comitato dei fondatori (da intendersi con modalità di adesione aperte, come soci della Fondazione), organo consultivo sulle materie di propria competenza. Si tratta peraltro, di soggetti che pagano una quota associativa paritaria di gran lunga inferiore a quanto loro stessi erano tenuti a versare con il vecchio Statuto. Altro organo statutario è il comitato scientifico, i cui componenti sono scelti tra esponenti del mondo accademico e della ricerca, in parte indicati dallo stesso comitato dei fondatori e in parte dal consiglio di amministrazione della Fondazione, a cui spetta, comunque, il potere di nomina. Con l'approvazione del nuovo Statuto appaiono, quindi, fortemente rafforzati i caratteri di terzietà e rilevanza pubblica della Fondazione, il cui finanziamento va ricercato in convenzioni e commesse di ricerca con e da parte di soggetti pubblici: Ministero dello sviluppo economico e altri Ministeri, Autorità indipendenti (segnatamente AGCOM), ed altri soggetti pubblici interessati. A seguito dell'approvazione del nuovo Statuto i professori Decina e Sassano hanno rassegnato le dimissioni dai lori rispettivi incarichi. Si è quindi proceduto, sulla base delle indicazioni statutarie, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che risulta composto da personalità di alto prestigio scientifico e professionale. Per quanto riguarda, in particolare, la notizia di stampa a cui l'interrogazione fa riferimento, sono i fatti stessi, a partire dal novembre 2008 sino ad oggi, a dimostrare come esse non avessero rispondenza con la realtà, dato che il dottor Di Luca non aveva allora, né ha oggi alcun incarico o rapporti di tipo professionale con la Fondazione Bordoni. Peraltro, il nuovo consiglio di amministrazione, tenuto conto in questa fase di avvio e sperimentazione del carattere di maggior rilievo che, con il nuovo Statuto, ha assunto la Fondazione, ha ritenuto opportuno concentrare tutte le responsabilità gestionali nella figura di Presidente. Pertanto, allo stato attuale, il direttore generale, pur statutariamente previsto, non è stato nominato e ciò anche in considerazione del fatto che le competenze più squisitamente tecniche vengono comunque assicurate dal direttore delle ricerche della Fondazione stessa. Per quanto attiene i criteri con cui si è proceduto alla nomina del consiglio di amministrazione, si è già ricordato come essi siano stati ispirati a professionalità e competenza indiscutibili e non vi sono ragioni che lasciano presupporre che, in futuro, in sede di nomina del direttore generale, non si tenga conto di tali criteri. Lo stesso consiglio ha poi eletto a presidente il dottor Enrico Manca, il cui profilo professionale è sembrato essere il più indicato in questo nuovo percorso della Fondazione Bordoni.

in cui si sottolinea ulteriormente il carattere di rilevanza pubblica della Fondazione Ugo Bordoni in relazione a previsti rapporti convenzionali e di ricerca da parte dei soggetti pubblici con la Fondazione stessa.

nota e stimata nel campo delle comunicazioni, rimane la domanda se fosse proprio necessario che il presidente avesse anche

in relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue. Il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 29 dicembre 2006, previo parere tecnico dell'ISPRA, ha accordato la deroga alla prescrizione tecnica che regola l'esercizio del deposito Avogadro. Ciò ha consentito il trasferimento temporaneo, per un periodo di tre anni, del solo combustibile irraggiato presente nella piscina di Eurex. Si è ritenuto «prioritario, imprescindibile e urgente l'adozione, da parte della Sogin S.p.A» delle azioni necessarie alla risoluzione della problematica della potenziale dispersione di acqua contaminata dalla piscina dell'impianto Eurex di Saluggia. Si è ritenuta, altresì, tale soluzione come l'unica praticabile, con maggiore celerità e, comunque, funzionale all'allontanamento definitivo del combustibile verso il riprocessamento all'estero. A seguito della citata deroga, il combustibile irraggiato dalla piscina Eurex di Saluggia è stato trasferito nel deposito Avogadro rendendo possibile lo svuotamento, la bonifica della piscina di stoccaggio dell'impianto Eurex e la risoluzione della problematica relativa alla potenziale dispersione di acqua contaminata. In relazione al riprocessamento in Francia del combustibile irraggiato italiano di cui all'Accordo intergovernativo del 24 novembre 2006 e dell'Addendum a tale accordo firmato, nel mese di maggio 2007, dal Ministro dello sviluppo economico *pro-tempore* con l'omologo Ministro francese, si fa presente che, a seguito di tale firma, Sogin ha perfezionato il contratto con la Società francese AREVA NC per il trasporto, il trattamento e il condizionamento, presso l'impianto francese di La Hague, del combustibile irraggiato italiano. Il programma generale di allontanamento del combustibile irraggiato, concordato dalla Sogin anche con la società AREVA, prevede l'allontanamento del combustibile stoccato negli impianti piemontesi mediante l'impiego

A tal proposito, si precisa che l'inizio delle spedizioni del combustibile ex Eurex, stoccato nel deposito Avogadro è, ad oggi, previsto a partire da marzo 2010 e l'allontanamento dello stesso dovrebbe completarsi, secondo le previsioni, entro giugno 2010. Successivamente, senza soluzione di continuità, sarà allontanato il combustibile ad ossido di uranio di Trino Vercellese ed il combustibile ad ossidi misti della centrale del Garigliano, stoccati anch'essi presso il deposito Avogadro. A conclusione dei trasporti dal deposito Avogadro, inizieranno i trasporti dalla centrale di Trino Vercellese che si concluderanno nel primo semestre del 2011. La tempistica per l'allontanamento del combustibile depositato in Avogadro è, dunque, condizionata dalla consegna dei relativi contenitori di trasporto. Riguardo alla solidificazione dei rifiuti radioattivi liquidi presenti in Eurex, che verrà effettuata, definitivamente, nell'impianto CEMEX, l'ISPRA ha fatto presente che, già dal 2001, sono stati presi provvedimenti diretti alla riduzione del rischio connesso alla loro presenza, tra i quali, il trasferimento, concluso il 26 novembre scorso, dei rifiuti liquidi a più elevata attività in nuovi serbatoi di stoccaggio posti in una struttura bunkerizzata denominata «Nuovo Parco Serbatoi». In merito al progetto dell'impianto per la solidificazione dei rifiuti radioattivi liquidi, CEMEX, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 19 settembre 2008, ha emanato il decreto di compatibilità ambientale (VIA) che è stato notificato a tutte le amministrazioni competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla sua realizzazione.

Per quanto attiene alla problematica relativa alla verifica e al controllo dell'infiltrazione della radioattività che potrebbe, eventualmente, essersi accumulata nel terreno e nelle falde freatiche, la campagna di monitoraggio idrogeologico e radiologico di tutta l'area interessata sarà proseguita dall'ISPRA, dalla Sogin, dall'Arpa Piemonte e dagli uffici tecnici delle Regione, della Provincia e dei Comuni coinvolti, ciascuno per quanto di competenza. Il Ministro dello sviluppo economico conferma la propria sensibilità al problema e si rende disponibile a svolgere ogni azione di competenza per il conseguimento dei comuni obiettivi di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente. Per quanto riguarda invece il controllo e la vigilanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sulle attività operative della Sogin Spa e di quanti operano nei siti nucleari l'ISPRA, competente in materia, ha fatto presente che, per l'intervento di bonifica della piscina Eurex, come per tutte le attività che comportano per i lavoratori il rischio di esposizioni alle radiazioni ionizzanti, la legge prescrive il rispetto di precisi limiti di dose (20 milliSievert all'anno), nonché l'adozione di provvedimenti protettivi di ottimizzazione atti a mantenere l'esposizione «al livello più basso ragionevolmente ottenibile». Con riguardo al 2007, anno in cui si sono svolte diverse attività all'interno del locale piscina, l'ISPRA ha precisato che le dosi da contaminazione interna dei lavoratori sono risultate tutte inferiori a un milliSievert (che è il limite di dose di legge per le persone), con sole due eccezioni di esposizioni totali annue leggermente superiori. Inoltre, ha riferito che nel 2008 è stata riscontrata una situazione sostanzialmente analoga.

per la sola individuazione delle procedure e della metodologia di selezione di un sito nazionale per la realizzazione di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi, comprendente anche il deposito nazionale. Il gruppo di lavoro Stato-Regioni, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, ha concluso i lavori il 25 settembre 2008, con l'elaborazione di un documento finale che delinea, oltre agli aspetti di carattere tecnico, le linee di un processo decisionale che vede il coinvolgimento delle Regioni e delle amministrazioni locali, in un percorso partecipativo basato sulle manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni locali.

problema che interessa non solo i Comuni sedi di impianti nucleari in via di disattivazione, ma anche settori diversi da quello dell'energia, come la ricerca, l'industria ed il settore ospedaliero.

mi sembra lasci insoddisfatto uno dei punti che nella mia interrogazione sollevavo e che il Sottosegretario ha affrontato al termine del suo intervento, quello cioè dell'individuazione del sito nazionale unico, definitivo per quanto riguarda lo smaltimento e lo stoccaggio delle scorie a bassa e media intensità, temporaneo per ciò che riguarda lo smaltimento e lo stoccaggio delle scorie ad alta intensità. Romani ha fatto riferimento al decreto Bersani del febbraio 2008, il quale prevedeva che entro l'anno scorso si sarebbe dovuta concludere l'istruttoria per l'individuazione del sito unico. L'istruttoria non si è conclusa, come abbiamo appena ascoltato, e quindi il problema che nel territorio di Saluggia e anche di Trino Vercellese, che è molto prossimo a Saluggia, crea grande preoccupazione è che la realizzazione dell'impianto Cemex per la cementificazione delle scorie liquide, a bassa, media ed alta intensità presenti nel sito di Saluggia avvenga in assenza dell'individuazione del sito unico nazionale. Come si sa, a Saluggia attualmente sono ospitati circa i tre quarti di tutte le scorie nucleari ad alta intensità presenti in Italia. Come si sa e come è certificato nello stesso parere di compatibilità ambientale che ha formato oggetto del decreto del settembre scorso relativo all'impianto Cemex, il sito di Saluggia è stato è stato dichiarato dai tecnici, in questa occasione ma anche in precedenti, inadatto a configurarsi come deposito stabile, se non definitivo,

dove provvisoriamente andrebbero stoccati i fusti cementificati dopo la cementificazione delle scorie liquide configura, in assenza dell'individuazione del sito nazionale, il rischio, che preoccupa molto quelle comunità, che Saluggia diventi, di fatto, il sito nazionale per lo stoccaggio delle scorie nucleari ad alta intensità, cioè di quelle più pericolose e dannose per la salute e decisamente incompatibili con le condizioni ambientali di quel territorio, in particolare con le sue condizioni geomorfologiche. Voglio ricordare che in passato ci sono già stati episodi, cui peraltro accennava il sottosegretario Romani, di infiltrazioni nelle falde acquifere dalla piscina della Eurex. Voglio ricordare che su quel territorio insiste un acquedotto che serve 300.000 cittadini di diverse province piemontesi. Insomma, quel territorio è sicuramente inadatto ad ospitare le scorie nucleari italiane ad alta intensità. In assenza dell'individuazione del deposito, credo davvero che la preoccupazione dei cittadini di Saluggia, di Trino Vercellese e di quell'area della Provincia di Vercelli sia fondata e che meriti risposte più puntuali da parte del Governo, tanto più che il Ministro dello sviluppo economico ha a più riprese dichiarato che in Italia ci sono moltissimi Comuni disposti ad ospitare il sito unico nazionale (anche se il nome di nessuno di questi è stato mai fatto). Quindi, si continua a camminare ed a procedere nell'incertezza; l'unica cosa certa è che a Saluggia sta per iniziare la realizzazione di un impianto per la cementificazione delle scorie che l'insieme di queste problematiche e preoccupazioni è ulteriormente rafforzato dalla scelta preannunciata dal Governo di riavviare in Italia la produzione di energia nucleare. È evidente il rischio che Saluggia diventi, di fatto, il sito stabile, permanente per lo smaltimento e lo stoccaggio delle scorie nucleari ad alta intensità, rischio ulteriormente accentuato dalla possibilità che l'Italia ricominci a produrre scorie nucleari ad alta intensità. Per queste ragioni

la legge n. 181 del 1989 fu approvata per far fronte alla grave crisi siderurgica degli anni Ottanta, con la finalità di promuovere nuove iniziative industriali, di rivitalizzare il sistema industriale locale e di creare nuova occupazione. L'applicazione delle agevolazioni, originariamente riservata esclusivamente ai progetti dì investimento che fossero stati realizzati nelle aree di crisi siderurgica specificatamente individuate, è stata poi estesa ad altre zone di crisi indipendentemente dalla vocazione siderurgica. La misura agevolativa è attualmente gestita da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (già Sviluppo Italia), ma fino al 1999 era gestita dalla SPI SpA, società oggetto di fusione per incorporazione in Sviluppo Italia. Relativamente agli incentivi percepiti dal gruppo Miroglio, si precisa che la SPI SpA ha deliberato, in data 13 luglio 1994, un intervento agevolativo, ai sensi della citata legge n. 181 del 1989, a favore della Filatura e Tessitura di Puglia SpA del gruppo Miroglio, finalizzato alla realizzazione di due siti produttivi localizzati nei comuni di Castellaneta e Ginosa, allo scopo di creare nell'area tarantina un polo tessile ad alta tecnologia per la produzione di filati e tessuti in fibre sintetiche ed artificiali. Il programma degli investimenti realizzato, pari a circa 77 milioni di euro, ha comportato l'erogazione di fondi pubblici complessivi pari a quasi 63 milioni di euro, (di cui circa 34,5 milioni a titolo di contributo a fondo perduto), con conseguente occupazione per 373 nuovi addetti. L'investimento è stato completato in data 27 marzo 1998 con la realizzazione dei due stabilimenti programmati, uno dedicato alla filatura e l'altro alla tessitura. Successivamente al primo intervento agevolato sopra illustrato, sono seguiti ulteriori due più ridotti programmi di ampliamento. Il primo, deliberato in data 20 marzo 1998, ha comportato investimenti per quasi 8 milioni di euro e un incremento di ulteriori 23 nuovi

ha riguardato invece il potenziamento di filo ritorto ed è stato realizzato interamente nello stabilimento di Ginosa, per una spesa di poco più di 6 milioni di euro. A favore del progetto sono stati erogati fondi pubblici pari a circa 3,8 milioni di euro milioni a titolo di contributo a fondo perduto). Tale investimento a comportato un ulteriore incremento occupazionale di 19 unità. Pertanto, i programmi di investimento a favore del gruppo Miroglio sono stati interamente realizzati con una spesa complessiva di 91 milioni di euro. complessiva dei progetti è stata pari a 413 nuovi posti di lavoro. La società ha usufruito di agevolazioni per complessivi 70 milioni di euro. Completato anche l'ultimo programma di investimenti, il gruppo Miroglio ha acquistato, in data 31 maggio 2001, la partecipazione detenuta dall'allora Sviluppo Italia (oggi Invitalia). Si fa presente, infine, che i contratti sottoscritti prevedono, a determinate condizioni, la revoca delle agevolazioni; tuttavia, gli obblighi contrattuali relativi anche all'ultimo intervento agevolato sono scaduti in data 26 gennaio 2007. Ciò premesso, relativamente alla domanda dell'interrogante circa la possibilità di verifica sul presunto trasferimento di alcuni macchinari ad altri stabilimenti del gruppo, si fa presente che il Ministero non ha più, attualmente, strumenti giuridici da poter porre in essere. Sono, comunque, allo studio sistemi giuridici e amministrativi più consoni a risolvere la problematica sollevata dall'interrogante. Relativamente, invece, al tavolo di trattative presso il Ministero dello sviluppo economico, numerose riunioni si sono svolte in tale sede, a seguito della volontà della Miroglio di dismettere gli impianti di Ginosa e Castellaneta. La proprietà, tuttavia, dava la propria disponibilità a mettere a disposizione i sopra citati stabilimenti per un nuovo imprenditore che avesse garantito la rioccupazione di tutti i dipendenti. Il Ministero, di conseguenza, si è impegnato a collaborare alla ricerca di un possibile investitore. Il 26 febbraio ultimo scorso, in una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato presentato il progetto per la reindustrializzazione dei due siti Miroglio. Tra le varie manifestazioni di interesse pervenute, è stata preferita quella del gruppo Intini di Bari, attivo nei settori delle costruzioni e della gestione dei rischi ambientali. L'investimento prevede anche la rioccupazione di tutte le unità lavorative, che sono circa 229. Gli occupati sono attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 mesi, per cessazione di attività, a decorrere da marzo 2009. Attualmente, si stanno predisponendo le misure per garantire la riqualificazione degli stessi, in quanto il gruppo Intini opera, come detto, in settori diversi da quello tessile.

migliore soddisfazione delle attese del territorio e dei lavoratori. Siamo quindi soddisfatti per quanto viene dichiarato. Attendiamo di poterci dichiarare in futuro pienamente soddisfatti se la riqualificazione del personale ci sarà, se l'azienda Intini si avvierà e se nel futuro, come aspetto generale, la ricerca del cosa, del come e del per chi e la verifica da parte delle strutture di vigilanza della giusta individuazione del cosa, del come e del per chi vengano

la trattativa tra il gruppo inglese Ineos ed il gruppo riconducibile alla finanziaria SAFI (facente capo al cavalier Sartor, un imprenditore veneto che, in controtendenza con quanto avvenuto negli anni più recenti, ha deciso di investire nella chimica) si è conclusa nelle passate settimane con la sottoscrizione di un contratto che prevede la cessione degli impianti di Marghera e dei siti sardi di Porto Torres ed Assemini. Con questo accordo SAFI si è sostituita ad Ineos nei preesistenti accordi sottoscritti con ENI presso il Ministero dello sviluppo economico, quegli accordi prevedevano l'ammodernamento e lo sviluppo degli impianti della filiera del cloro e cloroderivati. Il consolidamento della filiera del cloro a Porto Marghera ha, come conseguenza, un maggiore bilanciamento del *cracking* e, conseguentemente, il consolidamento della chimica di base nei siti padani di Mantova, Ravenna e Ferrara. Si ritiene, ora, necessario completare l'*iter* avviato con le intese citate. A questo proposito, sono in corso le trattative tra ENI e SAFI per la cessione degli impianti a monte di quelli già acquistati da Ineos. Si tratta, in particolare, delle saline di Contivecchi (Cagliari), degli impianti di cloro e dicloretano localizzati ad Assemini e a Marghera, dell'impianto di dicloretano e della costruzione del nuovo impianto di cloro celle a membrana che sarà realizzato con il concorso finanziario di ENI. dello sviluppo economico ha seguito e sta ancora seguendo con grande impegno ed attenzione, se positivamente conclusi, come si auspica, offrono prospettive di sviluppo ad una filiera strategica per il *made in Italy*, che conta 1.200 imprese di trasformazione a valle (nei settori dell'edilizia, degli elettrodomestici, telecomunicazioni, trasporti, mobile, eccetera) e che occupano circa 24.000 addetti, ai quali si aggiungono i 2.500 addetti che in modo diretto o attraverso l'indotto operano sugli impianti di produzione della materia prima. economico auspica che tutte le parti in causa, a partire da ENI, operino anche in queste ore per consentire la rapida conclusione dei negoziati e la conseguente sottoscrizione di accordi che rispondano agli interessi delle società in causa, ma anche agli interessi più generali del Paese.

prefettura, richiesto da tutte le istituzioni (Regione, Provincia, Comune), per sollecitare un impegno concreto e stringente e convocare in tempi urgentissimi un tavolo a Roma,

quel tavolo, utile a scongiurare un deterioramento pericoloso della situazione. È noto che a sostegno di questa vertenza più volte vi sono state azioni

dei lavoratori e delle maestranze degli stabilimenti di Porto Marghera, ha impedito che ciò avesse conseguenze ancora più gravi sul piano del governo di queste forme di protesta.

con un po' di buona volontà e con un impegno ulteriore sia possibile individuare una soluzione positiva nell'interesse di tutti e soprattutto di quelle migliaia di famiglie e di quegli imprenditori che vorrebbero davvero scommettere, non sulla scomparsa del polo di Porto Marghera e della lavorazione della chimica

di fronte ad una crisi dell'economia di dimensioni che non hanno precedenti, non esistono provvedimenti esaustivi e si devono porre in essere i possibili interventi sulla base della specificità delle diverse situazioni nazionali, dei vincoli di bilancio e della necessità di un coordinamento globale. In In questo quadro complessivo e in questa difficile realtà, questo Ministero sta sviluppando una possibile strategia al fine di fronteggiare il periodo di crisi con razionalità e per rendere il sistema economico più efficiente e competitivo. Tra le altre azioni di sviluppo intraprese si fa cenno all'istituzione del "tavolo di iniziative" per le piccole e medie imprese in attuazione dello *small business act* per il rilancio e la valorizzazione delle aziende di minore dimensione. In tale sede si analizzeranno tutte le tematiche del settore per formulare proposte concrete, atte alla semplificazione del lavoro e della burocrazia delle piccole e medie imprese.

Gli interventi sono assistiti dallo Stato, quale garante di ultima istanza, così che le piccole e medie imprese potranno fare affidamento su più consistenti volumi di finanziamento e ciò consentirà una forte accelerazione del processo di ripresa economica del Paese. all'istituzione del «tavolo sul settore della moda» al fine di salvaguardare un settore fondamentale del *made in Italy* e creare le condizioni per consentire alle imprese del settore di presentarsi più competitive sui mercati internazionali all'uscita della crisi. Tra le misure del tavolo si evidenziano il credito d'imposta per la realizzazione di campionari e collezioni; un bando *ad hoc* per progetti innovativi da finanziare con il fondo dell'innovazione tecnologica e le misure per promuovere prodotti certificati in termini di ecocompatibilità e sicurezza. al fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, cui possono accedere imprese di medie dimensioni con meno di 50 dipendenti e imprese di grandi dimensioni nella definizione di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 2003. Sulla specifica richiesta della crisi del gruppo Safilo, si premettono alcune informazioni generali su tale realtà industriale. Tale Gruppo, *leader* mondiale nel settore dell'occhialeria, con oltre 5.000 dipendenti, produce e commercializza, dal 1934, montature da vista, occhiali da sole e occhiali da sport. La struttura produttiva è articolata su quattro stabilimenti in Italia e due all'estero. In Italia, è presente in Veneto a Longarone,

La società ha progressivamente integrato il portafoglio di marchi di proprietà (Safilo, Carrera, Smith, Oxydo, Blue Bay) e soprattutto in licenza (Armani, Gucci, Valentino ed altri) e parallelamente ha aumentato la penetrazione commerciale in altri Paesi del mondo, in particolare negli Stati Uniti. La crisi finanziaria che ha portato, come detto, al rallentamento di quasi tutte le attività economiche e il settore specifico, al quale la società in questione appartiene, hanno sicuramente contribuito a generare le difficoltà che la Safilo sta attraversando. La crisi della Safilo, inizialmente seguita dalle istituzioni locali, ha assunto in questi giorni, una connotazione extraterritoriale. Il Ministro dello sviluppo economico, recatosi in Friuli-Venezia Giulia per una ricognizione delle aziende in crisi di quel territorio, ha annunciato l'istituzione di un tavolo di confronto nazionale, al fine di valutare il piano industriale dell'azienda. L'obiettivo è individuare un percorso che consenta di superare l'attuale momento di crisi e verificare ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva, possa continuare a operare nel territorio friulano e di evitare, ove possibile, tagli di personale. Gli uffici di questo Ministero hanno già contattato la proprietà, le rappresentanze dei lavoratori e le istituzioni locali, per convocare un tavolo che si terrà entro la prossima settimana. Tale incontro sarà utile per studiare, analizzare e definire i possibili interventi per il rilancio della società in questione.

insieme ad altri colleghi di maggioranza e di opposizione, ho presentato. Desidero farle rilevare, onorevole Romani, che questa è una crisi che riguarda certamente il territorio del Friuli-Venezia Giulia, ma che va valutata complessivamente ed è emblematica dei processi di riorganizzaizone del sistema produttivo italiano. Credo che il tavolo che lei oggi ha annunciato, e che si terrà la prossima settimana, dovrà affrontare alcuni nodi che, se non risolti, rischiano veramente di provocare

Se oggi c'è una crisi pesante di questo gruppo, la responsabilità è legata a tutta una serie di scelte sbagliate sul piano finanziario che si sono adottate negli ultimi anni, c'è stata una divisione tra i fratelli che avevano il controllo azionario della società, c'è stata una liquidazione di alcuni fratelli a carico dell'azienda con l'aumento pesantissimo dell'indebitamento, che oggi ha superato i 500 milioni di euro. Ma accanto a questa scelta, che ha appesantito la gestione finanziaria del gruppo, credo che le questioni di cui dobbiamo tener conto, e che mi auguro che il tavolo che il Ministero convocherà decida con grande chiarezza di affrontare, sono quelle legate al *made in Italy*. Non è possibile che alla fine si voglia decentrare in Cina, ad Hong Kong, noto paradiso fiscale, una parte della produzione che oggi è realizzata in Italia, in particolare nel Friuli-Venezia Giulia, solamente per cercare di aumentare i profitti in un campo dove dove la differenza di costo tra un occhiale realizzato in Italia e un occhiale realizzato in Cina è di pochi euro, ma i ricarichi sono pari a venti volte, cioè un occhiale che oggi costa dieci euro prodotto in Italia viene venduto a 200 euro quelli dei marchi che lei ha prima ricordato). È quindi inaccettabile per un Paese come il nostro che sostanzialmente vengano realizzati questi prodotti in Cina, con grande sfruttamento di manodopera a basso costo, che vengano riportati in Italia e venga poi apposto il marchio *made in Italy* quando si sa che sono prodotti in Cina. Pertanto, la prima azione che, in qualche modo, deve essere svolta è quella di tutela del *made in Italy*. Questo serve nel campo degli occhiali come nel complesso settore della moda. In secondo luogo, mi auguro che, in sede di tavolo, il Governo intervenga soprattutto nei confronti di Banca Intesa e di Unicredit, che sono i due istituti nazionali maggiormente esposti per alcune centinaia di milioni di euro, i quali oggi stanno cercando di recuperare un fondo americano per ricapitalizzare l'azienda, perché nel quadro della ricapitalizzazione della stessa favoriscano la rielaborazione di un progetto industriale che mantenga le unità produttive in Italia e, in e, in particolare, nel Friuli-Venezia Giulia. Questo intervento, su Banca Intesa, in particolare, è necessario anche alla luce del fatto che questi grandi istituti di credito hanno goduto, soprattutto negli ultimi tempi, dell'intervento dei Tremonti *bond*, in sostanza dell'azione del Governo per salvare il sistema creditizio italiano, e non possono poi scaricare poi scaricare i loro errori gestionali e finanziari su tutta una serie di aziende italiane (una di queste è proprio la Safilo), provocando disagi sociali e licenziamenti di migliaia di lavoratori. La terza grande questione è è la seguente: se non si dovesse riuscire a realizzare un'intesa legata alla ricapitalizzazione dell'azienda, quindi alla ridefinizione del nuovo piano industriale e ad un relativo blocco quantomeno del decentramento produttivo in Cina, credo che il Ministero dovrà affrontare - ci sono tutte

che il Sottosegretario ci ha comunicato che la prossima settimana verrà avviato questo tavolo. Mi auguro che il Governo, con la forza contrattuale che ha nei confronti dell'attuale proprietà e del sistema bancario, consenta un processo di salvaguardia dell'attività produttiva della Safilo nel nostro Paese e di tutela del *made in Italy*. Se riuscirà a raggiungere tali obiettivi dovremo sicuramente dargliene merito. In conclusione, aggiungo che lavoratori e sindacati si trovano in una situazione molto difficile. Per la prima volta sono anche scattate dinamiche di conflittualità tra le organizzazioni sindacali, nel senso che l'attuale gestione dell'azienda vorrebbe scaricare i tagli occupazionali - circa ottocento dipendenti - solo sul Friuli-Venezia Giulia. Questo